Grazie,

Signor Presidente, signor Ministro, una crescita considerevole del contenzioso tra Stato, Regioni e Province autonome. Dopo un primo tentativo di ridurre questo crescente contenzioso nella legislatura 2006-2008, successivamente, nelle ultime legislature le impugnative sono nuovamente aumentate. i dati quantitativi in merito alle impugnative fatte dai Governi Berlusconi e Monti nella XVI legislatura e dai Governi Letta e Renzi nella XVII legislatura.

Signor Presidente, signor Ministro, con riferimento alla facoltà del Governo di impugnare le leggi regionali davanti alla Corte costituzionale, si chiede di conoscere lo stato attuale del contenzioso, in particolare quali siano stati i motivi e le materie di legislazione di maggior conflitto.

ha portato alla nascita di un enorme contenzioso costituzionale tra lo Stato e le Regioni. Questo si è distribuito tra ricorsi proposti dallo Stato nei confronti delle Regioni, ma anche presentati dalle Regioni nei confronti di leggi dello Stato. Va detto subito che quella riforma della Costituzione fu portata avanti in modo autonomo dal centrosinistra, per iniziativa dell'allora presidente del Consiglio, Massimo D'Alema, e, dopo l'*iter* in Parlamento caratterizzato anche da forzature regolamentari, il 7 ottobre del 2001 fu approvato il *referendum* popolare confermativo, anche se con il voto del 34,4 cento degli italiani. Ci sembra di ripercorrere l'attuale cammino della riforma Boschi, che, andando nella direzione opposta a quella del 2001, cerca però di togliere poteri alle Regioni per riassegnarli allo Stato. Essa ha proceduto con forzature regolamentari ed è stata approvata a maggioranza, senza la condivisione più ampia che richiederebbe una legge costituzionale e, quindi, sarà sottoposta a *referendum*.

signor Ministro, come risulta dalla relazione del Presidente della Consulta sulla giurisprudenza costituzionale, anno 2015, i giudizi in via principale sono risultati 129: 55 proposti dallo Stato, 51 dalle Regioni e 23 dalle Province autonome. Le pronunce hanno prevalentemente avuto a oggetto discipline dello Stato, a fronte delle 39 che hanno riguardato leggi regionali. La Corte continua a segnalare la preponderanza di questioni promosse con riguardo al sistema costituzionale del riparto delle competenze legislative, specialmente per le materie di legislazione concorrente (e tra queste soprattutto il «coordinamento della finanza pubblica», il «governo del territorio» e la «tutela della salute»). Quantitativamente significative anche le censure proposte a proposito di funzioni amministrative degli enti territoriali e, soprattutto, della loro autonomia finanziaria e, ancora, del principio di leale collaborazione tra enti dello Stato. Si segnala l'impugnazione da parte di quattro Regioni ordinarie di numerose disposizioni (addirittura più di un terzo) dell'unico articolo della legge di riforma degli enti territoriali emanata nel 2014 (la cosiddetta legge Delrio). Appare evidente, dunque, il persistere di un modo di legiferare opportunisticamente scaltro, confusionario, raffazzonato, non conforme alla disciplina costituzionale vigente, nonostante il *dominus* assoluto del procedimento legislativo risulti il Governo con la decretazione d'urgenza. Quali intendimenti il Governo desidera assumere per supportare un processo legislativo parlamentare ordinario, volto ad annientare il perdurante contenzioso normativo tra Stato e Regioni?

Signor Presidente, signor Ministro, lo scorso febbraio la Commissione affari costituzionali, all'unanimità, ha conferito il mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea al fine dell'approvazione del nuovo testo unificato disegni di legge nn. 951 e 1082 (quest'ultimo a mia prima firma), recanti «Distacco del comune di Sappada dalla regione Veneto e sua aggregazione alla regione Friuli-Venezia Giulia». Il disegno di legge iscritto all'ordine del giorno è inspiegabilmente scomparso dal calendario d'Assemblea nella seduta del 16 marzo, ancor prima dell'inizio della discussione. Pur avendone chiesta la ricalendarizzazione, ad oggi nulla è dato sapere. È evidente quindi la volontà del Governo di opporsi alla definizione della vicenda. Infatti, finora non ci sono mai state esplicitate valide motivazioni a sostegno di tale comportamento per un provvedimento che poteva essere approvato anche in sede deliberante in Commissione stessa. Risale, infatti, al 2007 la delibera del Consiglio comunale di Sappada

oggi fornisca a me e ai sappadini le motivazioni che impediscono l'*iter* di un provvedimento atteso e le ragioni politiche che si celano dietro ad una scelta del Governo così incomprensibile e oscura. Chiedo inoltre con forza che il Governo riveda la decisione, porti a ricalendarizzare il provvedimento, ratificando immediatamente la volontà di autodeterminazione espressa nel rispetto della Costituzione. Grazie,

Negli ultimi anni la Regione Siciliana, in maniera particolare, è stata interessata da un grave contenzioso nei confronti dello Stato, principalmente a causa dell'infruttuoso funzionamento della Commissione paritetica Commissione paritetica per l'attuazione dello Statuto, che era prevista dall'articolo 43 dello stesso. Solo un esempio: negli ultimi tre anni una sola norma di attuazione è stata varata dalla Commissione paritetica e in tutto il 2016 la Commissione paritetica

le chiedo se il Governo intende per il futuro astenersi dal ricorrere ad aggiramenti delle previsioni dello Statuto che molto hanno mortificato quella Regione e quella popolazione e se intende rilanciare l'attività della Commissione paritetica attraverso atti formali e precisi, scongiurando, appunto, l'aggiramento della previsione statutaria che impone espressamente che le norme siano attuate attraverso la valutazione della Commissione. Signor Presidente, la riforma del Titolo V della Costituzione fu approvata frettolosamente nel 2001 dall'allora maggioranza di centrosinistra, si dice con l'obiettivo di guadagnare il consenso dell'elettorato della Lega, senza un'adeguata analisi delle sue implicazioni. Con la modifica del Titolo V della Costituzione si è aperta una stagione di riforme costituzionali. L'applicazione del nuovo Titolo V ha però creato problemi di interpretazione, aumentando il contenzioso tra Stato e Regioni con numerosi ricorsi alla Corte costituzionale. La riforma costituzionale propaganda - approvata adesso da questo Governo - cancella tutto il processo federalista che ha interessato negli ultimi vent'anni il nostro Paese, ridisegnando il sistema Stato, accentrando tutti i poteri e depotenziando i territori di propria iniziativa legislativa. La nostra riforma ideale vuole limitare la potestà legislativa esclusiva dello Stato alle sole materie necessarie a tutelare e garantire l'omogenea applicazione delle fondamentali funzioni dello Stato nazionale, concedendo alle Regioni l'autonomia legislativa su tutte le altre materie. Soltanto le amministrazioni più vicine ai cittadini possono comprendere appieno gli specifici bisogni e necessità della popolazione ed indirizzarvi in maniera razionale le risorse. Soltanto questa soluzione permette un vero risparmio sulla spesa pubblica. Questo la Lega lo ha proposto nella *devolution*, in cui si prevedeva un vero federalismo fiscale basato su un modello di riferimento virtuoso di fabbisogni e costi applicato in tutto il territorio nazionale, senza dimenticare le specificità di ogni Regione.

Bisogna intervenire al più presto. Questi stessi problemi ci sono sulla pianificazione territoriale, sulla finanza pubblica, sull'energia e le infrastrutture.

Come intende muoversi il Ministro per affrontare queste difficoltà, per chiarirle e superarle cercando di arrivare ad accordi per evitare localismi esasperati ma anche ingerenze eccessive e imposizioni del Governo nazionale, cioè in una parola, per essere virtuosi virtuosi e responsabili rispetto a questi problemi? Ci giochiamo una partita determinante e importante da qui al 2020. Se la perdiamo, se non ci confrontiamo seriamente, non so di cosa potremo parlare: saremo un Paese quasi da Terzo mondo.

Presidente, innanzitutto ringrazio molto per le osservazioni emerse da questo dibattito perché mi consentono di entrare nel dettaglio anche di un'evoluzione numerica

dalla consapevolezza, da parte degli enti locali, che i tavoli di confronto presso il Dipartimento per gli affari regionali erano tavoli proficui. un percorso che ha portato anche ad un rapporto di fiducia tra il Consiglio dei Ministri, il Dipartimento per gli affari regionali e gli enti locali, che in molte circostanze sfociato nel recepire degli impegni, meri impegni alla modifica di normative che non si ritenevano coerenti; poi stati mantenuti. Questo ha determinato un proficuo rapporto di collaborazione. Se nell'anno 2016 abbiamo raggiunto il numero minore di impugnative lo si deve a questo percorso. Il numero di atti che originariamente potevano destare perplessità è probabilmente rimasto inalterato, ma il percorso proficuo che si è generato ha subito delle modifiche. Una forma di negoziazione importante, una forma di collaborazione finalizzata al prevenire il più possibile i conflitti, è stata l'introduzione di strumenti di conciliazione tra Stato, Regioni e Province autonome, con particolare riguardo

ha operato una semplificazione e velocizzazione dei contatti tra amministratori centrali ed enti locali, i cui tempi tecnici più volte non hanno permesso di giungere a soluzioni condivise entro la scadenza dei sessanta giorni. Non dimentichiamo, infatti, che c'è un termine di scadenza che deve essere rispettato. Abbiamo cercato di velocizzare le procedure, giungendo molto spesso a degli accordi, a delle soluzioni tra le amministrazioni statali, che proponevano chiaramente delle impugnative per determinate ragioni,

in quanto l'insieme delle operazioni svolte dalla Corte a seguito dell'atto di promuovimento determina un indubbio dispendio di risorse. Impugnare per poi per poi fare marcia indietro sul ricorso, per effetto di un'attività istruttoria, è chiaramente un dispendio di risorse da parte della Corte costituzionale.

senatrice Orrù. Si osserva che nel corso degli anni si è assistito ad un incremento delle leggi regionali e provinciali sottoposte alla valutazione del Consiglio dei ministri. Se dal 2000 al 2011 la media non era stata superiore a 600 leggi annue, nel corso del 2012 sono state esaminate ben 702 leggi regionali, nel 2013 sono state rispettivamente 664 e 665. Allo stato, nel periodo tra gennaio e maggio del 2016 si è raggiunta la soglia delle 272 leggi esaminate. Rispondendo anche a quanto sostenuto dal senatore Morra, mentre nel periodo 2011-2012 si è assistito ad una crescita delle leggi impugnate rispetto al totale delle leggi esaminate, sia in termini assoluti (con un passaggio da 100 a 127), che in percentuale

predisposto l'iniziativa legislativa conseguente al *referendum*. Quanto ai quesiti del senatore le questioni prospettate circa la rinuncia a contenziosi e le erogazioni di risorse in favore della Regione Siciliana riguardano più specificatamente comportamenti propri del Governo nella sua interlocuzione con le Regioni. Analoghi accordi sono stati conclusi con altre autonomie speciali e hanno consentito l'erogazione di risorse certe da parte dello Stato a tutte le Regioni. Posso confermare di avere un grande rispetto e una grande attenzione per il ruolo della Commissione paritetica, che rimarrà centrale nell'esercizio delle sue competenze statutarie; anzi, se può essere utile un ruolo di propulsione e di attenzione sicuramente sarà mia attenzione svolgerlo. La senatrice Pelino ha posto le questioni relative all'eliminazione dell'incertezza normativa. Penso che la riforma costituzionale, che è stata

quanto, in questi anni di travagliata applicazione, la Corte costituzionale ha evidenziato. Quindi, sono convinto che ci sarà un contributo alla deflazione del carico. Ancora solo una risposta al senatore Centinaio: l'articolo 116 della Costituzione è un punto di riferimento fondamentale. Abbiamo ricevuto da parte della Regione Veneto la richiesta di avvio di una discussione e di un negoziato. È nostra intenzione confrontarci e avviarlo. Grazie, Signor Presidente, siamo molto soddisfatti della risposta del ministro Costa, perché dimostra come, con un continuo confronto tra

per cui, mancando ancora dei reali strumenti di collaborazione tra lo Stato e le Regioni, si scatenerebbe un nuovo contenzioso di natura nuova tra Regioni e Stato. Quindi, ci auguriamo una vittoria secca dei no al *referendum* di ottobre, che, oltre alla bocciatura della riforma Renzi-Boschi, dovrà guidare il prossimo Parlamento a correggere quegli errori della riforma del 2001 che hanno portato all'insorgere di questi contenziosi. Ministro, credo che non ci sia stata di fatto risposta a quanto ho domandato, perché di intendimenti, al di là di una generica volontà di ribadire un principio di collaborazione tra poteri e organi dello Stato, non si è parlato. Lei poi ha rimarcato come il contenzioso, in ultimo, sia stato in decisa attenuazione, ma ritenere che il 5 per cento, indicato per il 2016, considerando che non si sono conclusi ancora i primi cinque mesi dello stesso anno, Grazie, Ribadisco poi, in merito al futuro *referendum*, l'auspicio che possa essere chiaro a tutti in che direzione andare. Noi dobbiamo avere una qualità legislativa coerente con principi netti, chiari, di separazione di competenze. È vero che al livello formale qualcosa è stato fatto, però noi ci aspettiamo un aumento dei conflitti perché, soprattutto, per esempio... *(Il microfono

punto possiamo dire che sono lesi i diritti di una popolazione. Rispetto al discorso della Capigruppo, sa benissimo che c'è stata una richiesta congiunta; se poi c'è una volontà di maggioranza e di Governo che determina le scelte, credo non sia logico poi rimpallarsi quelle che sono chiare volontà di non affrontare il problema.

la ringrazio per la sua disponibilità ad attuare una formale sollecitazione nei confronti dalla Commissione paritetica. quando si riuscirà - spero prima o poi - ad evitare questo aggiramento delle previsioni statutarie, che fino ad oggi, sul piano di molti aspetti finanziari, è avvenuto, non sul tavolo istituzionale ma su altri tavoli. Signor Ministro, sono soddisfatto della risposta fornita. La speranza è che questo tavolo aperto con la Regione Veneto possa portare ad una maggiore autonomia e a maggior potere da parte della stessa Regione, sapendo benissimo che sarà solamente

la partita è nera per il Paese perché le risorse che abbiamo sono quelle; non ne abbiamo altre. Se non risolviamo questo problema e non lo affrontate come si deve, al di là di tutto, non so cosa dovremmo dire. Quando ho parlato di Terzo mondo

Signor Ministro, sostegno alle famiglie e natalità sono temi strettamente collegati. L'Italia è oggi in Europa il Paese a più bassa natalità e ciò - io credo - anche a fronte dei tagli che negli ultimi vent'anni tutti i Governi di centrodestra hanno hanno compiuto su politiche sociali, scuola e servizi per l'infanzia, indebolendo così - fino a farle scomparire - le politiche per la famiglia. Il Governo Renzi, invece, ha invertito tale atteggiamento ed ha compiuto scelte significative, a partire dalle politiche di conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare, la cui assenza troppo spesso ha costretto le donne e le coppie a scegliere tra Cito, ad esempio, la valorizzazione della maternità, anche con riferimento all'accesso e al mantenimento del lavoro, e la cancellazione delle dimissioni in bianco. Altrettanto importante è l'estensione della maternità retribuita anche alle lavoratrici autonome, nonché l'estensione dei congedi parentali con il relativo aumento dei figli nell'età dai tre agli otto anni, passando al *voucher* per le *baby sitter* fino a 600 euro al mese e al mantenimento del *bonus* bebè. Altrettanto importanti sono il cospicuo finanziamento per l'apertura di nuovi nidi e il riconoscimento del nido come diritto e non più come servizio a domanda individuale. Altrettanto importanti sono i sostegni economici a partire dal dal sostegno alle giovani coppie per quanto riguarda l'acquisto della prima casa e il relativo arredo. Altrettanto importante è il ripristino del fondo per le politiche sociali, passate da zero euro agli attuali 1,5 miliardi con la legge di stabilità del 2016. Essenziale è il fondo contro le povertà, dedicato alle famiglie con figli a carico. Finisco - ma potrei ancora fare molti esempi con l'inserimento nei livelli essenziali di assistenza della fecondazione assistita, perché sono ancora oggi troppe le coppie che desiderano figli, ma che non possono perché sterili. sterili. Nonostante le importanti scelte governative, permangono ancora grandi differenze tra Regione e Regione, le cui scelte, unitamente a quelle degli enti locali, determinano grandi disuguaglianze anche nelle politiche a sostegno della famiglia e della natalità. Sono pertanto a chiedere quali iniziative ella intenda adottare anche

è il Paese europeo a più bassa natalità; l'indice di natalità è tale da coprire appena la metà del numero dei morti che ci sono nel nostro Paese. o la nostra popolazione è destinata a decrescere fortemente oppure, come alcuni teorizzano, e come in ogni caso sta succedendo, si tratta di sostituire gli italiani con persone che vengono da fuori nei modi che ben sappiamo.

Vorrei dunque chiedere al Ministro che cosa concretamente intende fare il Governo, visto che nei primi due anni, ormai quasi due anni e mezzo di attività, per la famiglia ha ottenuto i risultati che ho descritto, oltre a spingere per tutte quelle leggi che tendono a disgregare la famiglia e a rendere più facile il divorzio che non il cambiamento di gestore telefonico.

per eliminare dal computo dell'ISEE le prestazioni legate alla disabilità, il Governo ha prodotto un emendamento che si rivela, ad avviso del Movimento 5 Stelle, un intervento tampone e inadeguato, che non rispetta appieno i dettami della sentenza, non diretto ad una riforma organica dell'indicatore e lesivo per talune categorie di disabili. Sono tre i nodi principali legati alla nuova configurazione dell'ISEE. In termini di calcolo della componente ISR dell'ISEE, viene eliminato con questo emendamento il precedente sistema di franchigia e viene inserito un sistema di calcolo fisso basato su un incremento di 0,5 alla scala di equivalenza ISEE. Questo fa sì che si favoriranno i nuclei familiari con redditi più alti a discapito di nuclei familiari a basso reddito, a cui invece si dovevano garantire maggiori tutele. Quindi l'emendamento non ripristina la normativa precedente e si rivela un *boomerang* non solo per le famiglie che hanno redditi minori, ma anche per i soggetti disabili gravi o non autosufficienti. fondamentale è quello legato al rimborso per le famiglie a cui sono state precluse agevolazioni legate all'utilizzo dell'ISEE, dichiarato illegittimo dalle sentenze. L'ultimo nodo sono le possibili conseguenze dell'erogazione delle prestazioni con questo nuovo indicatore e con la previsione di coperture non adeguate a coprire i costi aggiuntivi per gli enti. Le stesse amministrazioni per far fronte alle nuove spese moduleranno le soglie con un possibile aumento dei requisiti d'accesso, tant'è che all'interno del comma 3 avete inserito una dicitura del tipo: nel rispetto dei requisiti dei bilanci degli enti.

Sono noti gli effetti che questa dipendenza produce: la ludopatia è una vera e propria malattia e non un fenomeno sociale, che può condurre a rovesci finanziari, alla compromissione dei rapporti sociali, alla distruzione del proprio *habitat* familiare, al divorzio, alla perdita del lavoro, allo sviluppo di dipendenza da droghe o da alcol, fino al suicidio. Nonostante l'avvio di una campagna di mobilitazione su scala nazionale e la continua denuncia delle conseguenze disastrose di un tale piaga, dalla stampa si apprende di come l'Agenzia delle dogane e dei monopoli abbia emanato una circolare interpretativa con la quale, nella sostanza, a conti fatti, viene elevato il numero delle *slot machine* in Italia. Nonostante quanto disposto dalla legge di stabilità 2016, ovvero la riduzione delle suddette macchinette, nell'ordine del 30 per cento in quattro anni, di fatto gli apparecchi sono aumentati del 10 per cento in quattro mesi, ossia di 40.000 unità, passando da 378.000 a 418.000. Nello specifico, la legge di stabilità ha fissato un tetto ancorato al numero di *slot* esistenti al 31 luglio 2015 (378.000), oltre il quale viene precluso il rilascio di nuove autorizzazioni; tuttavia, in forza della suddetta ultima circolare dell'Agenzia, il tetto ora fa riferimento alle macchinette operanti al 31 dicembre 2015. Viene, infatti, precisato che tale numero è pari a 418.210 unità in quanto comprende sia gli apparecchi in esercizio sia quelli in magazzino sulla base delle liste fornite dai concessionari. La circolare aggiunge che la riduzione scatterà dal 1° gennaio 2017, ma intanto le concessioni scadute non saranno cancellate. Insomma, nel 2016 le 418.000 macchinette esistenti rimarranno al loro posto. Chiedo al Ministro come intende, nei limiti delle proprie attribuzioni, affrontare il problema del gioco d'azzardo, socialmente diffuso e praticato tramite macchinette, in termini di tutela della famiglia e quali sono le buone pratiche al fine di preservare la salute e l'economia delle famiglie, soprattutto alla luce della circolare dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di cui sopra.

la sperimentazione su scala nazionale dello *standard* *family audit*. Si tratta di uno strumento di *management* aziendale che consente all'azienda di porre il tema della conciliazione famiglia e lavoro al centro delle politiche aziendali. A livello nazionale sono ad oggi quasi 200 le organizzazioni che hanno conseguito questa certificazione familiare aziendale che evidenzia la strategia aziendale di conciliazione famiglia e lavoro. Di queste aziende circa il 50 per cento interessa il territorio della Provincia autonoma di Trento, mentre il restante 50 per cento è distribuito su tutte le altre Regioni italiane. Preso atto dei benefici positivi che questo processo genera per l'azienda in termini di flessibilità aziendale, motivazione dei dipendenti, riduzione degli straordinari e riduzione dei permessi per malattia figli e preso ancora atto che questo tipo di politiche consente di sostenere l'occupazione femminile e, quindi, la natalità, nonché di sviluppare un moderno sistema di *welfare* aziendale, si richiede al Ministro, visti gli indubbi benefici che esso genera e la sensibilità dimostrata in questo campo dal Governo e dal Ministro stesso, se intende procedere nel processo di diffusione nazionale dello *standard family audit*, già avviato favorevolmente in questi ultimi tre anni e come intende coinvolgere le Regioni e con quali finanziamenti. Io credo sia davvero una politica importante. *(AL-A (MpA))*. Signor Ministro, le dò alcuni numeri dell'ISTAT. Più di un italiano su quattro è a rischio povertà, è povero, nel senso che accusa la mancanza di risorse economiche adeguate che portano ad un accesso limitato ad ambiti sociali, come l'educazione, l'assistenza sanitaria, il lavoro, l'alloggio, la tecnologia, la vita politica e addirittura la vita sessuale. Sono proprio le famiglie numerose ad essere più vulnerabili

portando le famiglie a fare meno figli. La domanda è cosa intenda fare il Governo per cercare di dare un sostegno a queste famiglie più numerose, soprattutto per incentivare le famiglie a fare figli e a non limitarli in base al reddito.

quindi totalmente al di fuori dal contesto delle adozioni internazionali. Il Dipartimento antidroga è stato totalmente smantellato. Tutti i programmi di prevenzione, educazione e formazione nella scuola e per i genitori e di soccorso e aiuto sono scomparsi dal *radar*.

unioni civili. A questo punto c'è veramente da chiedersi quale sia il soggetto che secondo il Governo oggi è destinatario delle misure a sostegno della famiglia. Qual è il soggetto oggetto di queste

per dare ad ogni bambino il diritto di nascere da un padre e da una madre, il diritto di conoscere l'identità delle persone da cui nasce e di crescere anche con un padre e una madre.

la famiglia sia una società naturale fondata sul matrimonio), 30 e 31 della Costituzione enunciano in modo inequivocabile il regime preferenziale della famiglia quale nucleo fondamentale della società. Stando all'ultimo rapporto ISTAT, che ha diffuso gli indici demografici, le nascite in Italia continuano a calare: nel 2015 sono state 488.000. del numero dei figli per donna è di 1,35 al 2015 e si conferma questo *trend* in calo. La capacità dei genitori di investire sul futuro dei figli dipende da molti fattori, tra questi il loro stato occupazionale, di salute, il livello di istruzione raggiunto ed il sostegno nei compiti di cura che la comunità offre loro. La possibilità di disporre di competenze e risorse, non solo economiche, è essenziale, soprattutto nei primi anni di vita del bambino, quando l'offerta educativa e di relazione è decisiva per farne emergere le potenzialità. La denatalità in Europa è ormai un'emergenza. Entro il 2025 i primi Paesi europei - Italia, Spagna, Germania e Grecia - potrebbero sperimentare l'implosione demografica, ovvero la diminuzione effettiva della popolazione. non si risolverà con la legge che avete approvato ieri. È necessario affrontare in maniera sistematica la prima e più importante esigenza, rappresentata dall'avere una famiglia, cioè esistere. L'obiettivo principale deve essere quello di incentivare la natalità attraverso una serie di strumenti che intervengano nella fascia di età più delicata del bambino, ossia fino al compimento del terzo anno di età. delicata in termini educativi e di richiesta di attenzioni e cure, nonché in ragione della maggiore difficoltà di conciliare le esigenze familiari con quelle lavorative. È necessario conferire piena attuazione all'articolo 31 della Costituzione, che sancisce che «La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi (...)». A questo punto, vorremmo sapere quali politiche il Governo intende adottare per sostenere economicamente la famiglia e contrastare la piaga della denatalità. Non mi risponda ricordando la legge che avete approvato ieri.

vi ringrazio per questa occasione e per i ragionamenti e le considerazioni che sono state svolte. Lo faccio in modo non formale, perché

molte misure significative che, nel corso degli anni, sono state adottate proprio per raggiungere gli obiettivi e le finalità che oggi sono state evidenziati e declinati.

piuttosto frammentarie, frastagliate, disordinate e disorganiche. Faccio una riflessione da parlamentare, facendo anche un'autocritica perché in ogni legge di stabilità si è cercato di dare un contributo in termini costruttivi, che però non è mai stato organico e coerente con tutto il resto del percorso, anche precedente.

misure. Il DEF reca una indicazione di metodo che mi sono permesso di avanzare; sono contento che ci sia e

Il punto di riferimento, la classificazione normativa non è indifferente nell'attenzione che lo Stato ha nei confronti di una quindi questo è un aspetto di metodo che ritengo molto significativo. Io provengo dal settore della giustizia, di cui mi occupavo in precedenza, e quando si fa un testo unico anche in quel settore, significa che si vuole dare forte

centrato il tema della denatalità, che è il vero problema che affligge il nostro Paese. Lo indicano le statistiche, ma il dibattito parlamentare, quello tra i cittadini, i problemi dei cittadini ce lo fanno percepire al di là di ogni numero statistico. Il fatto che,

proprio per sostenere le famiglie con i figli e anche quelle con un figlio, atteso che il problema e la prospettiva di tante giovani coppie

per educare un figlio fino alla maggiore età, vediamo che sono molto pesanti e che normalmente il 35-40 per cento della spesa della famiglia è orientata all'educazione e al mantenimento del figlio.

conciliazione tra vita lavorativa ed educazione dei figli è stato evidenziato dai senatori Centinaio e Tarquinio. La legge n. 228 del 2012 ha introdotto la possibilità di fruire del congedo parentale anche su base oraria, demandando alla contrattazione collettiva le modalità applicative, a seconda delle esigenze del settore. Il *jobs act*, con le misure per la conciliazione delle esigenze di vita, cura e lavoro, ha introdotto significative modifiche volte a rendere più flessibile, anche nel pubblico impiego, l'utilizzo dei congedi parentali, aumentando l'arco di tempo in cui gli stessi possono essere fruiti.

Vi sono tante altre misure che sono finalizzate, chiaramente, a una flessibilità e a una conciliazione tra la vita lavorativa e l'educazione dei figli, perché ci sono tante mamme

La senatrice Mattesini ha evidenziato l'esigenza di avviare una ricognizione delle esperienze nei diversi territori sulle politiche di sostegno alla famiglia. Io sono d'accordo mia intenzione anche avviare - e lo dico in continuità e con rispetto per il lavoro svolto da chi mi ha preceduto (vedo qui il senatore Giovanardi) - l'aggiornamento dell'attuale piano nazionale della famiglia Senatore Giovanardi, rispondo soprattutto alla sua premessa. Ci sono delle articolazioni e delle attività organizzative nell'ambito delle deleghe assegnate che sono funzionali all'attività del Governo.

ai miei colleghi di Governo per arrivare a una disciplina organica. È una delega senza portafoglio, in quanto l'obiettivo è quello di far spendere agli altri colleghi del Governo, in modo organico ed efficace, a sostegno della famiglia, le risorse di loro competenza. Il senatore Barani ha posto delle questioni alle

deputati. Per finanziare questa delega si prevede la costituzione di un fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale di 600 milioni di euro per il 2016, incrementato, a partire dal 2017, con un miliardo all'anno. Vi è, poi, un'altra La senatrice Bencini ha posto la questione del gioco d'azzardo. Io ho evidenziato come si debba risolvere una contraddizione. Lo dico al di là della delega agli affari regionali, che mi porta, in Conferenza unificata, a presiedere un rapporto tra Governo ed enti locali. ed enti locali. Vi è una contraddizione tra uno Stato che non può prescindere da un'entrata e lo stesso Stato che avvia delle politiche per contrastare determinati rischi. Ho chiesto, proprio su questo tema, al Ministro dell'economia e delle finanze e al Ministro della salute di inserire un mio rappresentante un mio rappresentante nell'ambito dell'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave, un organismo istituto in attuazione della legge di stabilità 2015, proprio perché sono convinto che tale dipendenza incida pesantemente sulle relazioni familiari. Il senatore Panizza ha posto il tema del *family audit*, rispetto al quale sono particolarmente sensibile. Sono stato recentemente a Bari: Bari: la Regione Puglia ha recepito, in collaborazione con la Provincia di Trento (che è stata la Provincia in cui si è generata l'idea, sempre sostenuta dal Dipartimento della famiglia), il percorso del *family audit*. È un percorso molto significativo e qualificante anche di crescita delle imprese con determinate regole che siano vicine alle esigenze delle

che è oggetto del sindacato ispettivo, ripristinando un sistema di calcolo ISEE, limitatamente alla platea delle persone con disabilità, coincidente con quello previgente

avviare un rapporto, anche dialettico, sulle considerazioni che sono certamente da analizzare con attenzione, con il Ministro competente per materia che sicuramente, per quello che mi riguarda, potrà essere sensibilizzato. *(PD)*. Signor Ministro, sono soddisfatta della sua replica perché ha colto un passaggio importante. Nell'ottica della promozione e valorizzazione dell'importante lavoro che questo Governo ha fatto, giustamente si tratta di dargli ulteriormente forza proprio in questo elemento di raccordo. Lei lo ha chiamato

Credo anche che si debba lavorare con attenzione, e lei in parte lo ha sottolineato, sul fatto che oggi il Ministero è della famiglia ma la realtà è delle famiglie. Cito, senza altri appesantimenti di parole, l'ISTAT che ci dice

Signor Ministro, riconosco che lei riveste questa carica, e in particolare ha avuto la delega per la famiglia, da pochissimo tempo ma francamente non credo che dalle sue parole le famiglie italiane abbiano tratto

Resta il fatto che il Governo ha trovato i soldi per estendere il *bonus* bebè anche agli extracomunitari che di figli ne fanno già tantissimi, tant'è vero che nei loro Paesi sono troppi e vengono qui, ha trovato i soldi per dare 60.000 euro per ogni nuovo posto di lavoro alle aziende. Se si desse un terzo di quello che costa ogni immigrato all'Italia alle famiglie che fanno bambini, avremmo un *boom* demografico, e dovremmo fronteggiare una bella emergenza: quella di avere nuovi asili nido e nuove scuole. Purtroppo la politica del Governo, fino ad oggi, ha totalmente trascurato la famiglia.

da discutere come quella che proponiamo noi - il reddito di cittadinanza - che questa maggioranza non vuole discutere per chiari motivi, perché abolirebbe il voto di scambio politico-mafioso e il ricatto del lavoro. Per quanto riguarda l'ISEE, signor Ministro, certo che le interessa e interesserà certamente il Ministro competente, ma sicuramente anche lei. Le faccio un esempio che ha fatto sullo studio di HandyLex: una famiglia di tre componenti, composta cioè da due genitori con un figlio minore, che riceve l'indennità di accompagnamento e un reddito di 12.000 euro,

Signor Presidente, riprendo quello che ha detto il Ministro, cioè che lo Stato ricava una grande entrata dal gioco d'azzardo. Probabilmente tale entrata è più alta della spesa che poi affronta per curare le ludopatie. Ma purtroppo non viene quantizzato il danno sociale, patrimoniale e non patrimoniale del soggetto che cade in questa dipendenza. Mi fa piacere che nella legge di stabilità sia stato stabilito - scusate il gioco di parole - che venga nominata una figura competente, che lo affiancherà nel suo Ministero, per capire meglio

Signor Presidente, sono sicuramente soddisfatto per le parole con cui il Ministro ha espresso apprezzamento per il progetto dello *standard family audit* e anche per l'esperienza della nostra

ha detto il Ministro, soprattutto nella parte in cui ha fatto riferimento al fatto che, nel mezzo del cammin della sua vita, si era ritrovato in una selva oscura, come Vice Ministro della giustizia, dove le leggi si interpretavano e non si applicavano, mentre ora finalmente è ritornato a riveder le stelle, con la delega alla famiglia. Con questo testo unico sulla famiglia, magari diviso per il girone del Nord, del Centro e del Sud, dove c'è differenza di necessità e di esigenza, si può veramente riportare le famiglie a far figli. non è colpa del neo Ministro, tuttavia basterebbe fare le cose già indicate. Penso, ad esempio, al quoziente familiare e alla parametrazione del costo del servizio secondo il numero dei figli; è tutto scritto, ma nulla è stato fatto. Anzi, ieri è stato fatto il rovescio. A due uomini e a due donne che fanno un'unione civile si riconosce la reversibilità. un uomo e a una donna che vivono assieme per venti o trent'anni e che hanno dei figli non si riconosce né la reversibilità, né altri diritti che si danno alle coppie *gay*. È un Governo che si muove in direzione esattamente opposta a quelli che sono i diritti dalla famiglia prevista dalla Costituzione. me ne voglia il Ministro, ahimè non è colpa sua se per questo Governo la famiglia non è una priorità. Purtroppo si è preso un Ministero che magari il Presidente del Consiglio non ritiene prioritario, quello che è successo con la scuola in questi giorni. Sappiamo benissimo cosa sta succedendo: dieci milioni di italiani sotto la soglia di povertà non sono briciole. Sappiamo benissimo che questo Governo ha deciso di stanziare tre miliardi e 300 milioni per l'accoglienza di profughi profughi o finti profughi (non si è capito che cosa). Sappiamo benissimo che questo Governo, per combattere la denatalità, ha deciso di trasformare la famiglia tradizionale, la famiglia naturale, la famiglia prevista dall'articolo 29 della Costituzione e quindi concede agevolazioni a famiglie composte da uomo-uomo o donna-donna. Ci chiediamo come faccia. Visto che il Presidente del Consiglio è in grado di fare miracoli, ci chiediamo come faccia a combattere la denatalità

Il piano per i servizi socio-educativi per la prima infanzia, nel 2015, è stato rilanciato grazie a nuovi finanziamenti, pari a 100 milioni di euro, attualmente in fase di erogazione. Nel Documento di economia e finanza per il 2016 si prevede, entro il dicembre del 2016, il rifinanziamento del fondo per il rilancio del Piano di sviluppo dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, al fine di garantire politiche familiari che favoriscano la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Questa era la risposta specifica che dovevo